Nella seduta di oggi, dopo la discussione della ratifica tra Italia e Abu Dhabi su estradizione e mutua assistenza giudiziaria, si procederà alla votazione a scrutinio segreto, su liste bloccate, di nove membri effettivi e nove supplenti della delegazione italiana presso e nove supplenti della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. All'ordine del giorno di oggi è stata inoltre inserita la discussione del disegno di legge concernente la proroga del termine per la disciplina dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, che avrà luogo a partire dalle ore 17. Domani mattina, alle ore 9,30, si svolgerà il sindacato ispettivo per la durata di circa un'ora. Il resto della giornata sarà dedicato ai lavori delle Commissioni, salvo il *question time* alle ore 15. Saranno presenti i Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico, del lavoro e per gli affari regionali. Tenuto conto dello stato dell'esame in Commissione, la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge sullo sviluppo delle isole minori è rinviata alla prossima settimana. Nella seduta di martedì 9 ottobre sarà discussa la mozione n. 41, dei senatori Marcucci ed altri, e altre mozioni connesse, sui programmi di riqualificazione delle periferie. Restano confermati gli altri argomenti in calendario. La Conferenza dei Capigruppo ha altresì stabilito che, a seguito della remissione alla sede referente, la discussione dei disegni di legge

*Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018;* *Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)

*(FdI)*. Signor Presidente, con la ratifica di questi due Trattati conclusi con gli Emirati Arabi coloro che delinquono in Italia avranno un Paese in meno dove rifugiarsi nella speranza di sottrarsi alla giustizia. Per questa ragione, Fratelli d'Italia esprimerà un voto convintamente favorevole. In particolare, il trattato di estradizione risponde allo scopo di intensificare la cooperazione per contrastare più efficacemente la criminalità, tenendo conto che l'intensificarsi delle relazioni tra Italia e Emirati Arabi sul piano economico, finanziario e commerciale ha comportato anche lo sviluppo di fenomeni criminali che non possono rimanere senza un'adeguata risposta. Il Trattato di estradizione in esame disciplina, quindi, le procedure di consegna di persone ricercate perché sottoposte ad un procedimento penale o perché già condannate e che devono espiare la pena. In forza dell'articolo 2, comma 1, l'estradizione sarà sempre concessa a condizione che il fatto per cui si procede sia previsto come reato dai due ordinamenti (cosiddetto principio della doppia incriminazione). Allo stesso scopo del contrasto della criminalità è volto anche il Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale, che sancisce, in particolare, l'impegno dei due Stati a prestarsi reciprocamente la più ampia collaborazione in molteplici settori, tra cui la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione degli atti, la citazione di soggetti coinvolti in procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti e altri elementi di prova, l'informazione relativa ai conti bancari, l'assunzione di testimonianze e interrogatori di indagati e imputati, l'esperimento di perizie e consulenze, l'esecuzione di perquisizioni, sequestri e confische di cose pertinenti al reato. Infine, Infine, è previsto lo scambio di informazioni su procedimenti penali e condanne riportate dai cittadini dei due Paesi. In conclusione, come detto, con l'esecuzione di questi due Trattati, sarà più facile assicurare alla giustizia

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, dire che il Partito Democratico sostiene e voterà convintamente questo provvedimento perché in coerenza con iniziative già prese nella scorsa legislatura e frutto di un lavoro svolto da Governo e Parlamento, ma è meno pleonastico sottolineare il fatto che la convinzione sta nella consapevolezza che questo provvedimento è una parte molto importante della lotta contro la criminalità organizzata e tutte le mafie, un campo di battaglia che, per quanto ci riguarda, per non essere semplicemente evocato - vorrei dire retoricamente evocato - ma per essere effettivamente praticato, e con successo, deve avvalersi di un'analisi precisa e aggiornata e di provvedimenti conseguenti. Mi voglio riferire al fatto che stiamo intervenendo sulla dimensione internazionale del crimine organizzato e sull'adeguatezza degli strumenti per colpirlo. Parliamo, quindi, di un tema molto importante e quantomai attuale sul quale l'Italia

Mi piace ricordare, a questo riguardo, l'azione incessante intrapresa dalla Direzione della giustizia penale al fine di allargare la base giuridica convenzionale della cooperazione giudiziaria, un'azione che ha interessato decine di Paesi e diversi continenti: voglio solo ricordare i trattati già stipulati con Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Repubblica dominicana, Senegal, Nigeria, tutti rispondenti alla necessità di fondare su impegni vincolanti la collaborazione tra gli Stati nella lotta al crimine, uscendo dall'incerta e mutevole dimensione della cortesia internazionale a condizione di reciprocità. Non ci saranno più latitanti italiani che potranno confidare nel fatto di avere a poca distanza un facile e franco. Questo è il primo risultato concreto, che mette fine a una serie di tentativi che non avevano avuto successo per ottenere la consegna dei latitanti e conseguire conseguire l'efficacia e la credibilità delle decisioni del nostro sistema giustizia. Quando parliamo di effettività della pena, quando parliamo di impuniti o puniti, noi intendiamo questo: assicurare alla giustizia le persone che vengono condannate, in questo caso per gravi reati che colpiscono la comunità, in un quadro complessivo per colpire la criminalità organizzata. A questo riguardo, voglio ricordare che il quadro complessivo ha a che vedere con l'aggiornamento della platea dei reati (ne cito alcuni: caporalato, ecoreati e autoriciclaggio) nuovo codice antimafia e una riforma dei beni confiscati. Rivendicare questo lavoro svolto ovviamente non è piantare una bandierina perché

unito non solo in questo voto ma anche in futuro, deve impedire che si facciano passi indietro. Noi del Partito Democratico sicuramente ci metteremo di traverso per evitare che si facciano passi indietro. Mi sto riferendo Mi sto riferendo al fatto che siamo molto preoccupati in merito all'intenzione di questa maggioranza, manifestata nel contenuto del decreto sicurezza, di rendere possibile l'acquisto da parte dei privati dei beni confiscati alla mafia. mafia. Questo era un qualcosa che si era provato a fare nel 2008, ma che il ministro Maroni poi aveva corretto. aveva corretto. Già oggi è possibile ed è prevista la vendita dei beni confiscati, ma a certe precise condizioni: vendibili e acquisibili soltanto da enti pubblici. È inutile che si dica che si possono mettere cautele sui privati perché è evidente che, nel momento in cui sono accessibili ai privati, il prestanome è dietro l'angolo e quindi tutto ciò viene vanificato. Voglio a questo punto dire dire che non è un dettaglio tecnico. Qui c'è una differenza di impostazione e mi chiedo se nella maggioranza vi sia una condivisione di questa impostazione.

Se ci sono dei problemi, lo Stato non solo deve intervenire per risolverli, deve sostenere, essere presente e dare un contributo anche con innovazioni. Noi dei problemi delle aziende in crisi confiscate alla mafia ce ne siamo fatti carico. Siamo intervenuti nella scorsa legislatura e abbiamo provato, con successo, a risolvere questo problema perché

del MoVimento 5 Stelle, che sui beni comuni spesso siete intervenuti e intervenite, siete d'accordo su questa dismissione del bene comune? Siete d'accordo sul fatto che i beni confiscati perdano questo valore? Ne state discutendo? Noi su questo sicuramente non faremo fare passi indietro. Chiediamo anche a voi di discuterne e vogliamo vedere, alla prova dei fatti, come vi comporterete e come voterete su questo importante tema. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Non basta votare all'unanimità su un provvedimento e fare un po' di retorica sull'antimafia perché la mafia cambia; è cambiata negli ultimi vent'anni e, se la si vuole veramente combattere, bisogna essere presenti, impegnati e conseguenti.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, i due Trattati oggetto del presente disegno di legge di ratifica ed esecuzione rappresentano un significativo passo in avanti nei rapporti tra il nostro Paese e gli Emirati Arabi Uniti nell'ambito della cooperazione giudiziaria internazionale. L'estradizione obbligatoria, fermo il rifiuto obbligatorio nei casi in cui essa sia richiesta per reati punibili con la pena di morte, consentirà di rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, data anche la realtà sociale, caratterizzata da rapporti sempre più frequenti tra Italia ed Emirati Arabi nel settore economico, finanziario e commerciale. In questo senso, è dunque importante regolare in modo uniforme i procedimenti finalizzati alla consegna di persone sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena per i reati commessi. La reciproca assistenza giudiziaria in materia penale vuole invece favorire un miglioramento della cooperazione giudiziaria internazionale, attraverso lo scambio di informazioni e il ricorso a importanti strumenti quali la confisca dei beni. Questo è un fatto molto importante.

Presidente, concludo con questa importante affermazione: il Governo ha a cuore il rafforzamento della posizione dell'Italia all'estero e il suo ruolo fondamentale negli equilibri politici internazionali. La ratifica di questi due Trattati si pone in continuità con gli obiettivi dell'Esecutivo e in linea con il suo programma politico. Per tutti questi motivi, pertanto, il nostro voto sarà favorevole.

convintamente a favore della ratifica dei Trattati in esame in materia giudiziaria firmati con gli Emirati Arabi Uniti. Lo facciamo in sintonia con il voto che avevamo già espresso in 3a Commissione affari esteri, esteri, dove abbiamo avuto un ampio dibattito e dove alla fine il nostro Gruppo ha manifestato questa intenzione di voto favorevole sul provvedimento. Si tratta di accordi che puntano a implementare il contrasto alla criminalità e a migliorare la cooperazione giudiziaria di natura internazionale. Si intensificano - l'abbiamo sentito anche in quest'Aula poc'anzi - sempre di più i rapporti commerciali tra i nostri Paesi; quindi si adotta anche una più puntuale disciplina per regolare i rapporti in materia penale e di estradizione di eventuali criminali. Ovviamente sono previste, come evidenziano i princìpi fondamentali del diritto internazionale, condizioni di reciprocità, per cui il reato contestato deve essere previsto da entrambi gli ordinamenti. È inoltre prevista una stretta collaborazione per i reati di tipo fiscale, anche ove non siano esattamente sovrapponibili in entrambi gli ordinamenti. Nei Trattati sono altresì chiarite una serie di fattispecie ulteriori a garanzia dei sistemi giudiziari di entrambi gli Stati contraenti, è previsto il divieto di estradizione verso uno Stato terzo (un principio più che naturale), e altresì che lo Stato che concede l'estradizione venga puntualmente informato sull'esito del procedimento penale. Anche il Trattato di mutua assistenza in materia giudiziaria in materia penale firmato ad Abu Dhabi ha l'obiettivo condivisibile del contrasto alla criminalità. Insomma, con i Trattati che andiamo a ratificare dovremmo più leggere notizie di persone indagate, imputate o addirittura condannate che, in assenza di reciproca collaborazione tra i due Stati, possono girare indisturbate delle dorate spiagge del Golfo Persico, diventate a questo punto assolutamente impraticabili. Possiamo approvare questi accordi stando tranquilli,

estradizioni per motivi politici o per altri reati che non siano saldamente ancorati al nostro diritto positivo in materia penale. Pertanto, le garanzie del rispetto diritti fondamentali ci sono e ci rassicurano

va ad aggiungersi e sovente ad integrarsi con quella nostrana, animando la preoccupazione della nostra gente; pertanto, ogni strumento che possa limitarla è per noi il benvenuto. L'obiettivo deve essere L'obiettivo deve essere quello di creare un *network* globale di Paesi che si impegnano a sottoscrivere accordi di questo tipo. Quando la rete comprenderà tutti i Paesi si potrà avere una maggiore certezza che le garanzie espresse dallo Stato di diritto non possono essere aggirate. In questo senso consentitemi una digressione, rimanendo nel tema delle estradizioni. Prima di concludere rassegno solo una domanda al rappresentante del Governo: che fine ha fatto la pratica relativa Cesare Battisti, condannato all'ergastolo in via definitiva in Italia quale pluriomicida, al quale peraltro il Brasile ha revocato lo *status* di rifugiato,

colpito con un proiettile alla spina dorsale e rimasto su una sedia a rotelle, del commerciante Lino Sabbadin e dell'agente di polizia Andrea Campagna? Noi non li abbiamo dimenticati

delle vittime, soprattutto per la loro memoria, e dei familiari delle stesse. Con queste ultime considerazioni, signor Presidente, ribadisco il nostro plauso al disegno di legge in esame e il voto favorevole dei senatori del Gruppo di Forza Italia.

pochi minuti semplicemente per annunciare il voto ovviamente favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle sul provvedimento in esame che, oltre ad essere importante, è anche urgente perché, come abbiamo appreso durante il dibattito e anche dalle cronache, sono oltre

il nostro modo di stare all'estero e fare politica estera. Come abbiamo detto anche ieri pomeriggio, riteniamo sia importante dare un segnale

medie imprese che operano nel mondo. Dico questo perché molto spesso, soprattutto nella scorsa legislatura, abbiamo scoperto che

Grazie

Grazie

L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione di nove membri effettivi e nove supplenti della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Tale votazione avverrà, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento, a scrutinio segreto sulle seguenti liste di candidati formate su designazione dei Gruppi parlamentari. Membri effettivi, senatori: Bernini, Buccarella, Di Micco, Floris, Marinello, Perilli, Pirovano, Rampi e Vescovi. Membri supplenti, senatori: Fazzone, Ferrara, Guidolin, Laforgia, Marilotti, Rizzotti, Rojc, Rufa e Sbrana. I senatori favorevoli alle liste proposte voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si comporteranno di conseguenza. Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sulle

la coincidenza tra il numero delle tessere e i senatori

Presidente, chiedo scusa, ma il collega accanto alla senatrice Bernini non è presente e risulta aver votato a scrutinio segreto: questo non è accettabile. Mi stupisco della collega, che stimo per molte altre cose, ma in questa situazione rileva una caduta di stile e di e di conformità ai doveri etici minimi, anche di fronte ai ragazzi delle scuole. Non lo possiamo accettare.

proroga di un anno il termine per l'adozione, da parte del Governo, di uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive al codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174. La proroga del termine si rende necessaria al fine di poter emanare decreti integrativi e correttivi adeguatamente meditati. In simili materie il cosiddetto diritto vivente costituisce, come noto, un criterio guida per la correzione di tali normative e provvedimenti. L'anno in più che si sottopone all'attenzione di quest'Assemblea ha dunque esclusivamente lo scopo di consentire di realizzare una normazione in linea con le esigenze che si sono manifestate durante l'applicazione concreta delle disposizioni in oggetto.

Grazie

pubblica amministrazione, e anche del decreto legislativo 26 agosto del 2016, n. 179, che ha riguardato il riordino dei giudizi di fronte alla Corte dei conti. la maggioranza e il Governo ci chiedono di avere più tempo per procedere all'emanazione di eventuali disposizioni integrative e correttive. Non vediamo ragioni per opporci a tale richiesta, ma annunciamo alla maggioranza e all'Assemblea che ovviamente saremo molto vigili e attenti per quanto riguarda i contenuti effettivi che

Grazie

Presidente, intervengo per richiamare all'attenzione del Ministro delle infrastrutture una mia iniziativa di sindacato ispettivo, la riguardante la mancata definizione della copertura finanziaria in seguito ad attività di espropriazione per la realizzazione dell'autostrada senza pedaggio Chieti-Pescara. Sono circa trent'anni che quest'opera è stata definita e una norma del nostro ordinamento prevede che, quanto alla definizione dei contenziosi riferiti a tale genere d'infrastruttura,

C'è un ritardo da parte del Ministero delle infrastrutture, nella direzione generale competente, per corrispondere la copertura finanziaria necessaria a superare l'attuale situazione di contenzioso,

sulle iniziative assunte o da assumere per portare a conclusione giuridica il *dossier* di quest'infrastruttura fondamentale, che consentirebbe lo spostamento di oltre un milione di persone sull'area urbana Chieti-Pescara. La ringrazio, signor Presidente, per la sollecitudine con la quale il Ministro assicurerà la sua presenza in Aula.

Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo in quest'Aula per rilanciare il grido di dolore che dalla mia Regione, l'Abruzzo, tanti cittadini stanno inutilmente elevando nel silenzio assordante della politica e di chi per troppo tempo li ha male amministrati. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Intervengo per denunciare in Parlamento il delitto perfetto che si sta consumando su di loro, popolo inquinato che con grandi speranze ma inutilmente ha atteso giustizia per uno dei più gravi episodi di inquinamento ambientali mai registrati non solo in Italia ma anche in Europa. Venerdì scorso, onorevoli colleghi, la IV sezione penale della Cassazione ha messo la parola fine sul processo per il disastro ambientale di Bussi sul Tirino. Oggetto dell'accertamento l'ipotesi di commissione dei reati di avvelenamento delle acque sotterranee e di disastro ambientale in capo a diversi *manager* e responsabili della sicurezza Montedison, proprietaria del sito per gran parte del secolo scorso. Una vicenda giudiziaria che inizia più di dieci anni fa quando, il 12 marzo 2017, venne posta sotto sequestro la discarica Tre Monti a Bussi, un'area boscata proprio davanti a un grande petrolchimico per anni nella gestione di società del gruppo Montedison, scoperta dal Corpo forestale dello Stato guidato dal compianto comandante Guido Conti. stata una lunghissima udienza preliminare, diversi incidenti di percorso e finanche la ricusazione del presidente della corte d'assise di Chieti, in prima battuta individuato per aver pronunciato, nel corso di un'intervista ad un giornale, una frase, una semplice frase: faremo giustizia per il territorio. La sentenza di assoluzione in primo grado ha negato la stessa esistenza dell'avvelenamento e ha dichiarato prescritto il disastro, considerandolo colposo. In secondo secondo grado la decisione è stata ribaltata con una pronuncia in cui la corte d'assise d'appello ha riconosciuto l'esistenza dell'avvelenamento delle falde acquifere, seppure prescritto, ed ha condannato una parte degli imputati per disastro aggravato. Quei giudici hanno ritenuto fondate le domande risarcitorie dello Stato, della Regione Abruzzo, degli enti locali e delle associazioni ambientalistiche, condannandoli al pagamento di provvisionali. A distanza di più di un anno e mezzo, la Cassazione ha azzerato quel risultato, annullando senza rinvio la sentenza aquilana; una sentenza che è risultata pesantemente manomessa a causa del comportamento del giudice Romandini che sui giudici popolari chiamati a decidere insinuò il dubbio che in caso di condanna di quei responsabili avrebbero potuto essere chiamati a ripagare il danno, il tutto con il sottofondo di una misteriosa tangente che, come sa un illustre componente di quest'Aula, il senatore D'Alfonso, sarebbe occorsa per orientare il processo. A questo punto stupisce che la Cassazione abbia accolto le ragioni di quella sentenza così pesantemente messa in dubbio per le cose dette ed abbia fatto proprie le ragioni di una sentenza, che a questo punto non possiamo che definire manipolata, per azzerare un processo nel quale la Cassazione dice che c'è inquinamento, ci sono i responsabili, c'è la popolazione di tutta la Val Pescara che continua - a causa di questi pozzi inquinati

che, per un episodio così grave di inquinamento, gli inquinatori la fanno franca e forse i cittadini italiani, non sono gli abruzzesi, dovranno pagare le spese per disinquinare quel sito. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. L'unica speranza di giustizia, a questo punto (e noi ci contiamo), è che il Ministro dell'ambiente si metta in campo per trovare la soluzione a questo problema, affinché siano gli autori dell'inquinamento a pagare e non più il popolo inquinato, che continua a rischiare la propria salute e a dover mettere le mani ancora nelle proprie tasche per pagare i danni ambientali

Signor Presidente, onorevoli senatori, oggi sul Colle San Marco, sopra Ascoli Piceno, si è celebrato il 75° anniversario dell'inizio della lotta di Liberazione. Il Colle San Marco sovrasta Ascoli Piceno e, per la sua posizione strategica, fu scelto immediatamente come punto di raccolta e di lotta dagli antifascisti. Quelle lotte hanno segnato per sempre il mio territorio e anche le nostre memorie. Gli scontri che si sono susseguiti negli ultimi anni di guerra fra le correnti partigiane e le schiere nazi-fasciste iniziarono nel Piceno subito dopo l'armistizio e culminarono il 3 ottobre del 1943 quando, sul Colle San Marco, furono uccisi dai nazisti i partigiani del luogo che, tra i primi in Italia, erano insorti per la libertà della nostra Patria. Questi eventi hanno permesso sia alla Provincia sia alla città di Ascoli Piceno di insignirsi della medaglia d'oro al valor militare per l'attività partigiana. Mi sia permesso in questa sede quindi ricordare il 3 ottobre di settantacinque anni fa, perché esso rappresenta un giorno di tristezza per tutti noi, ma anche di profondo coraggio. La commemorazione di episodi così violenti deve servire essenzialmente come collante fra le generazioni, per evidenziare l'importanza della memoria storica in quanto utile anche per la comprensione del presente e per le scelte che facciamo immaginando il futuro. Essa va coltivata come monito per non ricadere negli stessi tragici errori e per tenere bene a mente il vero significato e i veri valori che hanno poi portato alla nascita dell'Europa. Infatti, in un momento particolare come quello che stiamo vivendo, in cui l'Europa ci appare purtroppo una rigida ragioniera imprigionata nei propri conti e poco attenta alle richieste dei cittadini, ricordare significa invece riesumare l'idea e la consapevolezza che l'Europa stessa nasce dalla visione di un futuro pacifico e libero da conflitti cruenti, basato sulla democrazia e sull'uguaglianza tra i popoli e le nazioni, e su quei valori di collaborazione e ascolto reciproco che devono essere rispettati, oggi più che mai, in tutti i settori e in tutti i campi, proprio perché il prezzo della loro conquista è stato troppo alto da dimenticare.